L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca: «Votazione per l'elezione di due componenti del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA». Per questa votazione ciascun senatore riceverà una scheda sulla quale indicherà, ai sensi dell'articolo 63, comma 15, lettera del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, un solo nominativo tra coloro che hanno presentato la propria candidatura nell'ambito della procedura di selezione prevista dal comma 16 del medesimo articolo 63 del decreto legislativo n. 208 del 2021, il cui *curriculum* è pubblicato nel sito Internet del Senato. Saranno proclamati eletti i due candidati che otterranno il maggior numero di voti. Dopo la chiama, che avverrà in ordine alfabetico, le urne resteranno aperte fino alle ore 13, mentre l'Assemblea proseguirà nell'esame del successivo punto all'ordine del giorno. Dichiaro aperta la votazione e invito il senatore Segretario a procedere all'appello

Onorevoli colleghi, poiché le Commissioni riunite 5a e 6a non hanno terminato l'esame del decreto-legge recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico, passiamo direttamente al punto successivo dell'ordine del giorno.

Presidente, gentili senatori, rispondo all'interrogazione 3-00806, presentata dalla senatrice Rando. Desidero innanzitutto rappresentare che il Ministero è attivamente impegnato nella diffusione della cultura della sicurezza all'interno delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo primario di garantire alle studentesse e agli studenti spazi sicuri e idonei all'apprendimento, alla socializzazione e alla convivenza civile. Nella convinzione che il tema della sicurezza nelle scuole non debba limitarsi alla celebrazione di una giornata a essa dedicata, ma debba costituire un impegno costante, il Ministero, attraverso campagne di informazione e attività di formazione sulla gestione dei rischi, condivisione di buone pratiche, collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali, continua a ribadire che la sicurezza a scuola è un diritto inalienabile per gli studenti, il personale scolastico e le famiglie. A tal proposito, segnalo che si sta procedendo al rinnovo del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il dipartimento della Protezione civile, denominato «Azioni di collaborazione per la sicurezza nelle scuole», la cui scadenza è prevista per il prossimo novembre. Inoltre, in vista dell'approssimarsi della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, fissata come di consueto per il 22 novembre, il Ministero si sta attivando per il rinnovo dell'accordo di collaborazione con Cittadinanza attiva. Mi preme sottolineare che, proprio in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, ma non solo in tale occasione, il Ministero è impegnato nel sensibilizzare e sostenere le istituzioni scolastiche affinché promuovano iniziative didattiche e formative e formative sul tema. Il Ministero ha inoltre fornito supporto al Ministero per la protezione civile e le politiche del mare nella distribuzione del fumetto «L'attimo decisivo - La virgola» nelle scuole secondarie di primo e secondo grado situate nella zona rossa dei Campi Flegrei, attività da noi promossa anche attraverso il sito istituzionale. Tra le iniziative di rilievo, segnalo l'adesione di questo Dicastero alla campagna nazionale «Io non rischio», che prevede percorsi esperienziali e attività laboratoriali, gestite dai volontari della Protezione civile, sui temi inerenti ai rischi naturali e alle norme di comportamento, già avviata in collaborazione con alcuni uffici scolastici regionali. Nell'ambito delle attività previste in collaborazione col dipartimento della Protezione civile, desidero inoltre ricordare i campi scuola «Anch'io sono la Protezione civile», lo sviluppo di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento sul tema, nonché la partecipazione al progetto «Edurisk» e ad altri progetti di rilevanza internazionale. La collaborazione tra il Ministero e il dipartimento della Protezione civile si è ulteriormente concretizzata nella condivisione dei dati del Sistema nazionale dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, che ha permesso l'elaborazione di nuove mappe ai fini della valutazione del rischio sismico. Infine, per quanto riguarda l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, desidero rassicurare che il Ministero si sta impegnando per convocare la prossima riunione proprio in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Concludo assicurando che è di vivo interesse del Ministero, come testimoniato dalla sintetica illustrazione fin qui fornita, promuovere e rafforzare ogni iniziativa volta alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi, affinché la sicurezza sia davvero un diritto.

per sensibilizzare sulla sicurezza nelle scuole. Questa celebrazione, per esempio, l'anno scorso non ha visto la presenza del Ministero e Grazie quando abbiamo presentato questa interrogazione non risultava nessuna circolare e nessun tipo di informazione rispetto a questo. Io le voglio credere sulla parola, però la Giornata è alle porte e, di norma, la si prepara con un certo margine di tempo. C'è un altro tema, signora Sottosegretaria, che a noi sta particolarmente a cuore. È la convocazione dell'Osservatorio sull'edilizia scolastica. La legge relativa è del 1996;

nel ventennio in cui l'Osservatorio, nonostante fosse previsto per legge, non è stato mai contattato, perché l'Osservatorio serve, insieme all'anagrafe, non solo per attuare quella mappatura e per verificare lo stato delle nostre scuole. Lei ha fatto bene a ricordare Cittadinanzattiva,

senza aggiornare l'anagrafe secondo i criteri necessari, noi ci ritroviamo a non sapere quali sono gli interventi che devono essere fatti. Signora Sottosegretaria, aggiungo che, purtroppo, anche le risorse per l'edilizia scolastica non sono così

che i risultati in questi due anni sono questi. Non si vuol attuare una misura perché fatta dai Governi precedenti e quindi si creano problemi nella continuità, anche programmatica, che serve ai nostri enti locali, dalle Regioni ai Comuni. Spesso, Spesso, i nostri Comuni vengono lasciati soli e poi si trovano di fronte a situazioni che capitano e non sanno perché. Siccome a tutti noi sta a cuore la spero davvero che alla giornata del 22 novembre il Ministero dia il rilievo dovuto, perché è un momento di sensibilizzazione che serve a quello. ai bambini nella formazione sulla sicurezza, che è importantissima, non serve a loro. Serve a tutti noi per ricordarci che di edilizia scolastica dobbiamo continuare a parlare. Spero che, a questo punto, l'Osservatorio venga convocato al più presto.

è doveroso precisare che i decreti ministeriali che regolano le procedure concorsuali ordinarie per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché della scuola dell'infanzia e primaria, stabiliscono che i bandi di concorso possono prevedere, in caso di esiguo numero di posti disponibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali. Inoltre, la stessa disposizione prevede che, con decreto del Direttore generale per il personale scolastico, possano essere disposte ulteriori aggregazioni, anche nel caso di esiguo numero di aspiranti. Sulla base della disciplina vigente, il Ministero con i decreti direttoriali 89 e 90 del 18 gennaio 2024, 2024, relativi rispettivamente alla scuola dell'infanzia e primaria, alla scuola secondaria di primo e secondo grado, ha disposto le aggregazioni delle procedure concorsuali, sia in caso di esiguo numero di posti disponibili in una determinata Regione, sia in caso di esiguo numero di aspiranti che hanno presentato domanda per una determinata Regione. Sulla base di quanto esposto, il Ministero, nel predisporre le aggregazioni secondo le modalità sopraindicate, ha comunque cercato di tutelare al meglio la posizione di coloro che hanno presentato domanda per la Regione Sardegna. In particolare, con riferimento all'aggregazione legata al numero esiguo di posti disponibili per la scuola dell'infanzia e primaria, il bando ha previsto aggregazioni territoriali soltanto per i posti di sostegno, designando l'USR Toscana come ufficio responsabile della procedura concorsuale. Per quanto riguarda, invece, la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono stati previsti accorpamenti solo per cinquantuno classi di concorso e tipologie di posto. Questa tipologia di aggregazione ha avuto, peraltro, un impatto relativamente limitato sulla Regione Sardegna rispetto ad altre Regioni per le quali sono stati previsti un maggior numero di accorpamenti. A titolo esemplificativo, per la Regione Sicilia sono state previste aggregazioni per cinquantacinque classi di concorso e tipologie, di cui sei presentavano un numero di posti superiore a Inoltre, a livello nazionale, dall'esame dei dati risulta che circa 109.000 candidati non sosterranno la prova orale nella Regione di destinazione. Di questi, solo il 2,91 per cento ha presentato domanda per la Regione Sardegna. Questo dato assume rilevanza se posto a confronto, ad esempio, con la Regione Sicilia e la Regione Campania, dove i candidati che sosterranno la prova orale in una Regione diversa da quella per cui hanno presentato domanda sono rispettivamente pari al 10,38 e al 16,23 per cento. Infine, si sottolinea che, al fine di salvaguardare nel miglior modo possibile gli aspiranti docenti che sosterranno la prova orale in una Regione diversa da quella per cui hanno presentato domanda, entrambi i bandi di concorso prevedano che la traccia da sviluppare per la lezione simulata venga estratta dal candidato ventiquattr'ore prima dell'orario programmato per la prova. A tutela del candidato che non possa essere presente all'orario previsto per l'estrazione, la Commissione procederà in ogni caso all'estrazione della traccia e ne darà comunicazione al candidato tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Grazie Signor Presidente, signora Sottosegretaria, mi sembra che questa sia una risposta molto burocratica e formale. Mi rendo conto che lei ha riportato le valutazioni sulla base delle quali

città non vicine a Roma o a Milano, dalla Sardegna non c'è continuità territoriale e si devono spendere tanti soldi. Lei mi dirà che ciò vale anche per la Sicilia e io credo che anche per questa Regione si debba prevedere un trattamento specifico e differente. In più, ci sono persone che magari possono sostenere più prove e quindi devono viaggiare tra diverse altre Regioni. Sappiamo che

sarebbe giusto che voi assumiate l'impegno di affrontare un nodo che riguarda anche altre condizioni. Faccio riferimento a una questione che ho trattato mesi fa, in interrogazioni rispetto alle quali non ho ancora avuto una risposta (ma speriamo sempre che in futuro la diate) sul sul dimensionamento scolastico, su cui abbiamo presentato anche degli emendamenti. La Sardegna è una Regione che ha una specificità, ovvero una densità di popolazione molto ridotta, e sottoporre alla stessa regola la Sardegna e la Lombardia della senatrice Malpezzi non ha molto senso, perché si applica l'autonomia scolastica scolastica in una località rispetto alla quale gli istituti distano decine e decine di chilometri, tante attività che si organizzano nell'ambito degli istituti stessi si svolgeranno con maggiore difficoltà e tutto questo allontana gli studenti della scuola, ritarda necessità di favorire tutto ciò che può migliorare una condizione che - lo ripeto - se guardiamo i numeri è davvero drammatica. L'abbandono scolastico e il livello di istruzione sono un dramma per le Regioni meno sviluppate d'Italia e la Sardegna è tra queste. A mio avviso, sia per attuare la Costituzione sia per garantire l'eguaglianza dei cittadini e la coesione territoriale e sociale che i provvedimenti sull'autonomia differenziata stanno in in realtà rallentando e sostanzialmente distruggendo, sarebbe bene che il Governo si ravvedesse e stabilisse che almeno per il futuro sia garantita l'uguaglianza sostanziale delle persone che vogliono e possono accedere a un posto stabile da docente, di cui c'è tanto bisogno per loro e per gli studenti, in particolare nella mia Regione, ma credo in tutta l'Italia.

merito*. Signor Presidente, il tema del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è di forte interesse per il Ministero dell'istruzione e del merito, il quale ha adottato numerose iniziative per prevenire e contrastare tali fenomeni, in particolare all'interno delle istituzioni scolastiche. Desidero innanzitutto sottolineare l'importanza dell'educazione civica nel contrasto al bullismo. Le nuove linee guida adottate con decreto ministeriale n. 183 del 7 settembre scorso si configurano, infatti, come strumento di supporto e sostegno ai docenti, specialmente di fronte gravi emergenze educative e sociali del nostro tempo, tra le quali rientra di certo anche l'aumento di atti di bullismo e di cyberbullismo. Nel nucleo delle nuove linee guida, che include l'educazione alla legalità intesa come promozione del rispetto delle norme per il benessere di tutti i cittadini, rientra anche l'educazione contro ogni forma di discriminazione e bullismo. Per il contrasto al fenomeno del bullismo abbiamo, inoltre, previsto una revisione della disciplina sulla valutazione del comportamento che sta per divenire legge proprio in questi giorni. Con questa riforma il bullo dovrà sempre di più assumersi la responsabilità delle proprie azioni svolte in ambito scolastico. Rispetto alla precedente normativa che prevedeva la sospensione a casa, la nuova legge favorirà la permanenza a scuola con approfondimenti e attività di cittadinanza solidale. Ricordo inoltre che la legge n. 70 del 2024, che modifica la legge n. 71 del 2017, ha ampliato il campo di applicazione della stessa, estendendo la prevenzione e il contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e al contrasto anche del bullismo. L'accento è posto su azioni preventive, su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia in qualità di vittime sia di responsabili di illeciti, privilegiando interventi di carattere formativo ed educativo. La suddetta legge prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisca un tavolo permanente di monitoraggio composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti del settore. Ancora, al fine di rafforzare l'impegno verso un'azione educativa mirata alla cultura del rispetto, all'educazione alla relazione, al contrasto alla violenza maschile sulle donne, il Ministero ha emanato la direttiva «Educare alle relazioni». Infine, nell'ambito delle azioni di educazione per un uso corretto e consapevole della Rete e delle tecnologie digitali, il progetto «Safer internet center-Generazioni connesse» rappresenta una delle iniziative più significative del Ministero. Questo progetto ha sviluppato un percorso di formazione rivolto ai docenti, finalizzato alla realizzazione di un documento programmatico interno all'istituto. Tale documento è fondamentale per programmare o aggiornare le attività di cittadinanza digitale, riconoscere, gestire e monitorare episodi legati a un utilizzo scorretto delle tecnologie digitali e per individuare azioni didattiche di prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che diventano quindi parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa. Al quadro sin qui delineato aggiungo con orgoglio che è di pochi giorni fa la notizia che per la prima volta una scuola italiana è tra le tre finaliste del premio per la migliore scuola al mondo per un progetto contro il bullismo, confermando che le iniziative da noi intraprese sono giuste e proficue. Concludo confidando di aver dato prova che le azioni illustrate costituiscono iniziative concrete che sono state svolte da questo Governo nel forte convincimento di dover intervenire a monte per prevenire i fenomeni del bullismo e i casi, come quelli richiamati nel presente atto ispettivo, che denotano una preoccupante perdita di valore delle relazioni tra i giovani.

agiate soprattutto per reprimere. Oggi leggiamo su tutti i giornali di queste nuove norme, a cui ha fatto cenno anche lei, sul voto di condotta e sulle sospensioni. È un po' la traslazione - mi perdoni - della politica criminale del Governo, infatti quando agite sul codice penale, lo fate aumentando le pene e i reati. Ce n'è una lunga lista nel

signora Sottosegretaria, se lo lasci dire da un signore ormai di una certa età, che però è stato un adolescente gay in un liceo del Mezzogiorno d'Italia negli anni Ottanta: i ragazzi sono meravigliosi perché sono tutti diversi gli uni dagli altri, perché sono in un certo senso non conformi, perché c'è sempre qualcosa per cui si può essere bullizzati - puoi avere gli occhiali, puoi avere una taglia un po' più grande di quella desiderabile secondo certi schemi, puoi avere la pelle di un altro colore

si decidesse a prendersi la responsabilità di parlare di rispetto reciproco, di accettazione reciproca, di spiegare che non esistono dei modelli preordinati, che non è vero come dicono alcuni esponenti - ogni riferimento al generale Vannacci è puramente casuale che tutto ciò che non rientra nella maggioranza non è normale. La scuola dovrebbe occuparsi anche di raccontare che il *range* della normalità

però, questa responsabilità dovrebbe prendersela e non dovrebbe poi urlare, come per esempio si fa normalmente, contro la dottrina *gender*. Dire, per esempio, a una ragazzina che vuole fare l'ingegnere meccanico che va bene o dire a un ragazzino che vuole fare il ballerino classico che va bene servirebbe moltissimo a prevenire questo tipo di fenomeni e questo non significa dire loro che possono cambiare sesso, ma significa dire che ogni ragazzo e ogni ragazza ha diritto a compiere il percorso verso le proprie aspirazioni aspirazioni e i propri sogni anche se non sono propriamente quelli della maggioranza dei loro amici e delle loro amiche di scuola, e questo non lo si fa. Bisognerebbe, per esempio, anche approvare leggi dello Stato volte a passare il messaggio che avere modelli di vita, di affettività o un colore un colore della pelle che non sono quelli della maggioranza va bene. Se noi avessimo una legge che dice che i ragazzi che sono nati qui sono italiani qui sono italiani o che le due mamme di quella nostra compagna di scuola sono sposate come le mamme e i papà degli altri, passeremmo dei modelli di inclusione potentissimi e nelle scuole

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento, invito tre senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede e al computo dei voti La seduta è sospesa.

*(Applausi).* Non c'è molta gente, ma chi c'è ha applaudito. Credo che l'applauso sia anche perché è stato rispettato il senso di un eletto di maggioranza e un eletto di opposizione, al di là del numero dei votanti. I lavori dell'Assemblea riprenderanno alle ore 15 con il question time con i ministri Calderone e Zangrillo. *(La seduta, sospesa

il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

come lei ha più volte affermato, nel 2023 nel settore pubblico sono state reclutate oltre 170.000 persone, lo stesso numero viene replicato quest'anno ed è in progetto anche per il 2025. Si tratta di un piano di assunzioni estremamente importante, anche in considerazione del fatto che nei prossimi dieci anni andrà in pensione all'incirca un milione di dipendenti pubblici. È quindi assolutamente necessario sostenere le amministrazioni con nuovo personale, anche in considerazione degli impegni stringenti previsti dal PNRR. In questo percorso di importante rinnovo dei dipendenti della pubblica amministrazione è fondamentale approntare misure per renderla attrattiva nei confronti delle giovani generazioni e anche nei confronti di quei giovani quei giovani che definiamo i giovani cervelli, che troppe volte ci lasciamo sfuggire verso altri Paesi. Tra l'altro, signor Ministro, le devo fare i complimenti per la campagna di comunicazione del suo Ministero, perché ha centrato il punto: i giovani non sono più tanto interessati al posto fisso, ma sicuramente al posto "figo", perché vogliono essere valorizzati,

non delle migliori: tra il 2009 e il 2020 la pubblica amministrazione ha perso 300.000 persone per effetto del blocco del *turnover*; l'età media dei dipendenti pubblici è passata da quarantaquattro a cinquant'anni; ora siamo di fronte a una transizione demografica veramente significativa: un milione di persone nei prossimi cinque o sei anni. Abbiamo però invertito la rotta e avviato una nuova stagione di assunzioni. Grazie alla completa digitalizzazione delle procedure concorsuali, oggi, con il portale inPA, siamo passati da tempo medio della durata delle procedure concorsuali a centottanta. Lei ricordava che abbiamo inserito 670.000 persone nel 2023 e altrettanto faremo nei prossimi tre anni. anni. Per dirvi che non stiamo parlando soltanto di sogni o di aspirazioni, ma di realtà, da gennaio ad agosto di quest'anno abbiamo pubblicato 13.200 bandi, abbiamo bandito 288.000 posizioni e abbiamo ottenuto 2,1 milioni di candidature. Questo significa che un po' di attrattività la pubblica amministrazione ancora ce l'ha. Abbiamo messo a terra iniziative finora sconosciute al pubblico impiego per attrarre i giovani e cercare di migliorare il mix generazionale: lo abbiamo fatto con il contratto di apprendistato per i neolaureati e con il contratto di formazione e lavoro per i ragazzi di età inferiore ai ventiquattro anni. I ragazzi vengono selezionati e hanno poi la possibilità, al termine del contratto, di essere confermati a tempo indeterminato. Da quest'anno, il 2024, abbiamo inserito altre due iniziative, i tirocini e i dottorati, per consentire a chi sta completando gli studi universitari o si è appena laureato di scoprire le dimensioni della pubblica amministrazione. Nello specifico, abbiamo attivato 300 tirocini curriculari della durata di sei mesi per un valore di 600 euro mensili e 20 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca della durata di tre anni, con una retribuzione di 30.000 euro all'anno. Stiamo poi registrando anche anche importanti e significativi miglioramenti sul fronte delle competenze. Anche il tema della formazione era un'altra delle criticità della nostra organizzazione. Alla fine del 2022, il tempo medio dedicato alla formazione dei dipendenti pubblici non raggiungeva le sette ore all'anno. Oggi, con il potenziamento del nostro portale digitale Syllabus, le nostre persone già nel 2024 sfiorano mediamente i tre giorni all'anno di attività formativa. L'obiettivo evidentemente è quello di puntare ai migliori talenti a cui noi dobbiamo offrire - come lei ricordava, senatore Rosso - prospettive di crescita e di valorizzazione, dal punto di vista non solo economico, ma anche professionale. Ed è questo il motivo per il quale molto presto, credo entro la fine dell'anno, presenterò un disegno di legge per un nuovo sistema di assegnazione di obiettivi e di valutazione della *performance* a cui legare la carriera delle nostre persone. Per concludere, modalità e tempi di accesso rapidi, nonché sviluppo delle competenze, a cui dobbiamo aggiungere anche sistemi gestionali a onor del mondo, quindi volti a premiare il merito, sono gli elementi e le carte su cui dobbiamo puntare per vincere la scommessa del futuro: una pubblica amministrazione all'altezza dei suoi compiti.

perché emerge che stiamo lavorando nella giusta direzione, con le nuove assunzioni (facendo la somma, ci avviciniamo a quasi un milione di posti di lavoro attrattivo per i giovani), la formazione continua (che porta alla crescita personale

ma anche altre cose che sta portando avanti lei con il suo Ministero, come le semplificazioni e la digitalizzazione. Questi sono grandi temi, utili per rendere finalmente efficace ed efficiente la pubblica amministrazione, e lei,

in una formula, con il Governo Meloni questo non è più un Paese per giovani e vi dimostro perché. Ci sono dati drammatici sull'occupazione, davvero allarmanti, che preoccupano e che non ci fanno percepire speranza nel nostro Paese, ne sono altri molto brutti sul piano degli stipendi per gli *under* 35: il 43 per cento percepisce uno stipendio mensile inferiore a 1.000 euro. Abbiamo dati che ci indicano che i Millennials, ma anche la generazione Z, guadagnano meno rispetto ai propri genitori, mentre secondo dati molti recenti il costo della vita continua ad aumentare. Dal 2022 al 2023 100.000 giovani italiani si sono trasferiti all'estero. Le azioni che questo Governo ha messo in atto per recuperare talenti e cervelli dall'estero sono state però penalizzanti e hanno messo in discussione anche quella positiva impostazione che aveva voluto il Governo Renzi nel passato, producendo così un effetto negativo su queste cifre. È del tutto evidente che un Paese che vuole provare a giocare la carta dell'innovazione e la sfida della modernità, come primissimo obiettivo deve avere quello di creare un ambiente giusto

è stato messo in atto ed è davvero una grande delusione. Ho sentito spesso parlare di famiglia da parte di questo Governo e ricordo che la famiglia sono innanzitutto i figli

sollevata dai senatori interroganti è certamente di rilievo, dal momento che ci si riferisce al tema delle retribuzioni e dell'inserimento lavorativo dei giovani, sul quale il il Ministero del lavoro sta ponendo la massima attenzione. In questa direzione credo vadano le misure già introdotte, come ad esempio, gli sgravi contributivi e gli specifici incentivi che hanno rimesso in moto il circuito produttivo, favorendo assunzioni e contratti stabili. Questo è l'ultimo indicatore. Il nostro mercato del lavoro ci restituisce un aumento dell'occupazione stabile anche nella fascia giovanile. In particolare, mi riferisco certamente all'occupazione di giovani e donne: abbiamo messo in campo azioni concrete per il riconoscimento del diritto alla riqualificazione delle competenze e per la garanzia dell'occupabilità sul posto di lavoro e nelle transizioni da lavoro a lavoro. Basti ricordare che, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Piano nuove competenze ha l'obiettivo di rafforzare la formazione professionale e innalzare il livello delle competenze delle persone in cerca di occupazione e sostenere le transizioni dei lavoratori. decreto coesione abbiamo introdotto meccanismi qualitativi per la valutazione della formazione finanziata, legandone l'efficacia e l'effettivo ingresso al lavoro dei fruitori della formazione. Stiamo facendo un lavoro apposito affinché la formazione finanziata sia valutata in termini di efficacia legata all'ingresso lavorativo. Credo inoltre che per i giovani l'accrescimento delle competenze ai fini del miglioramento dell'occupabilità sia fondamentale. In questo senso, ricordo il rafforzamento dell'offerta dei percorsi di formazione duale e la recente riforma del sistema di formazione professionale, che ha creato una maggiore coerenza dei percorsi di formazione di secondo grado. Al riguardo, voglio ricordare che il decreto coesione incentiva l'assunzione a tempo indeterminato di giovani privi di occupazione stabile. Sto parlando del nuovo *bonus* giovani, che riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono giovani *under* 35 con contratto di lavoro

con una dotazione complessiva di 800 milioni di euro, e incentivi all'autoimpiego nei settori strategici e per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, con una dotazione di 239 milioni. Ribadisco che, nell'ambito delle valutazioni sulla prossima legge di bilancio, resta saldo l'impegno del Governo a prorogare la riduzione del cuneo contributivo e fiscale. Sono inoltre allo studio di questo Ministero ulteriori misure per dare impulso all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, a favore *in primis* di giovani e donne, delle quali si sta verificando la compatibilità con le politiche di bilancio. Ribadisco pertanto che il percorso da promuovere è certamente quello di un lavoro equo, dignitoso e che possa saldare le esigenze delle diverse generazioni. Su questo assicuro i senatori interroganti la massima attenzione per quanto riguarda il Ministero

allarmanti sul tema dell'occupazione: ha fatto bene perché non avrebbe avuto argomenti per contrastare i dati che ho citato. Devo dire che apprezzo l'onestà intellettuale, ma apprezzo meno il lungo elenco di azioni che evidentemente, visti i dati, non stanno dando i risultati che servono a questo Paese e ai nostri giovani. Bisognerebbe cominciare a tracciare una linea, perché non è passato un giorno da quando il Governo migliore di questa Repubblica si è insediato di fronte ai cittadini: cominciano a essere due anni e in questo arco di tempo i risultati sono quelli che ho dato io, non il lungo elenco che la Ministra ha voluto fornire a tutti noi, perché in quel lungo elenco di risultati non ce ne sono stati, non ne sono stati prodotti. Faccio alcuni esempi: l'intervento sulla questione del costo dei libri di testo è un grande tema che riguarda le famiglie; interventi per quanto riguarda gli sgravi sulla formazione, sulle certificazioni sulla lingua straniera sarebbero un grande aiuto alle famiglie. Perché avete voluto eliminare la 18app, cioè uno dei pochi interventi che consegnava ai nostri giovani autonomia nella formazione e nell'acquisto di libri, anche di carattere universitario? Vi siete riempiti la bocca il tema degli affitti per gli universitari, ma non avete intrapreso un'azione che vada in quella direzione. Oggi ci dite che probabilmente riuscirete a confermare il cuneo fiscale. Vi lanciamo una sfida: noi abbiamo bisogno non solo di confermare il cuneo fiscale, come già Draghi aveva fatto, ma di avere un intervento specifico, duraturo, costante sulle giovani generazioni, altrimenti questo Paese non avrà speranza. mi spiace moltissimo prendere atto che anche un Ministro tecnico come lei abbia ceduto notevolmente all'impostazione della demagogia politica, perché in quel lungo elenco di effetti e di risultati per i nostri ragazzi non ce ne sono.

Presidente, signora Ministra, il settore della pubblica amministrazione ha subito significativi tagli lineari e indiscriminati, con ripetute revisioni della spesa pubblica in Italia. Questi interventi includono il decreto-legge n. 138 del 2011, introdotto per affrontare l'instabilità finanziaria, e il decreto legge n. 201 del 2011, noto come salva Italia, che ha introdotto la riforma Fornero del sistema pensionistico. Inoltre, ci sono state altre misure successive, come il decreto-legge n. 95 del 2012 e il decreto-legge n. 101 del 2013 per la razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni. Si consideri inoltre che la disciplina di erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR) e del trattamento di fine servizio (TFS), modificata ai sensi del combinato disposto dei provvedimenti che ora ho citato, rappresenta oggi, di fatto, un elemento di oggettiva disparità tra lavoratori del settore pubblico e del settore privato e che la regolamentazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori del settore pubblico presenta disparità appunto rispetto a quello del settore privato. Nel pubblico impiego, infatti, i tempi di attesa per il pagamento del trattamento variano da un minimo di 105 giorni ad oltre due anni a seconda della causa di cessazione del lavoro. Al contrario, nel settore privato i tempi di attesa per il TFR sono definiti dalla contrattazione collettiva, con una scadenza che va da un massimo di 30 giorni nel terziario a 45 giorni nel commercio. L'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisce poi le modalità di erogazione dei fondi: un solo pagamento annuale se l'importo è fino a 50.000 euro, due pagamenti annuali se l'importo è tra 50.000 e 100.000 euro, tre pagamenti annuali se l'importo è oltre 100.000 euro. Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza n. 130 del 23 giugno 2023, ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio sulla disparità di trattamento tra TFR e TFS. Questa questione era emersa da un ricorso di un dipendente pubblico che richiedeva il pagamento immediato del TFS ritenendo il pagamento rateale lesivo dell'articolo 36 della Costituzione. La Corte ha dichiarato incostituzionale il rinvio del pagamento dei trattamenti di fine servizio, affermando che questi fanno parte della retribuzione e devono essere erogati in modo tempestivo. Nonostante ciò, l'INPS continua a versare il TFR seguendo criteri ritenuti illegittimi dalla sentenza senza fornire spiegazioni. Si chiede pertanto di sapere quali iniziative ancora di carattere normativo il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare attuazione alle decisioni della Corte costituzionale e quali siano le motivazioni per cui ancora perduri la disparità di trattamento.

della disparità di trattamento nell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto o servizio tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato. In merito all'interrogazione oggetto di questa discussione, è opportuno evidenziare che nel settore pubblico i termini di pagamento delle prestazioni di TFS e TFR sono differenziati in base alla causale di cessazione dell'iscritto, come diceva il senatore interrogante. Come è noto, questa differenziazione deriva dalla disciplina contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 97, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, sulla quale è intervenuta la Corte costituzionale, richiamata dagli interroganti, sebbene esclusivamente in riferimento alla disposizione che differisce di dodici mesi la liquidazione di questi emolumenti in caso di ordinaria cessazione dal servizio. Come la stessa Consulta ha osservato, sebbene il differimento possa incidere sulla funzione previdenziale propria delle predette prestazioni, non si può non considerare che tali prestazioni costituiscono un aggregato della spesa pubblica di parte corrente particolarmente rilevante. Per questa ragione si rappresenta che, nelle more di un intervento normativo di più ampio respiro, il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS ha già adottato una deliberazione, la n. 2 del 2024, con la quale a legislazione vigente ha inteso adottare un piano di azione concreto volto a superare, da un lato, eventuali ritardi dovuti alla mancanza di risorse umane e materiali per l'elaborazione delle istanze e, dall'altro, a introdurre le più idonee misure normative per garantire un'adeguata tutela alla platea dei lavoratori interessati. Occorre invero considerare che nel solo 2023 sono state liquidate 624.000 pratiche, le quali, al netto di un congruo numero di importo modesto legato alle liquidazioni delle supplenze brevi del comparto istruzione, impattano in modo ben più che significativo sulle risorse pubbliche disponibili, circostanza che rende imprescindibile un intervento non solo complessivo, ma soprattutto coordinato con tutti i Ministeri interessati. Il tema è pertanto all'attenzione del Ministero, il quale ha avviato, in necessaria sinergia con il Ministero dell'economia e delle finanze, le necessarie procedure istruttorie al fine di addivenire a un risultato in linea con quanto evidenziato dalla Consulta, nel rispetto delle inderogabili esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

soddisfatti della sua risposta. Inoltre, le sottolineo che questo Governo ha una bella gatta da pelare che si aggiunge ad altre, ovviamente, visto che siamo anche in procedura di infrazione. Solo il prossimo anno si prevede infatti che vadano in pensione 150.000 dipendenti pubblici, calcolando una media di 70.000 euro ciascuno di buonuscita si arriva ad una spesa cospicua fino a 10,5 miliardi di euro che, come abbiamo appreso adesso, non avete intenzione di gestire visto che vale quasi una mezza finanziaria. A ciò però si aggiunge anche la mancata rivalutazione delle indennità di buonuscita dei lavoratori postali per circa un miliardo. Buonuscita dei postali che non è rivalutata dal 28 febbraio 1998 e coinvolge 200.000 postali. Io credo che sia giunto il momento - e il nostro MoVimento 5 Stelle lo sottolinea con forza - di porre fine a questo sequestro per dipendenti pubblici. È un sequestro illegittimo delle liquidazioni dei dipendenti pubblici. Ribadiamo con forza a questo Governo che il differimento del pagamento della liquidazione dei dipendenti pubblici è anticostituzionale dal momento che contrasta con il principio della giusta retribuzione contenuta nell'articolo 36 della Costituzione.

Signor Presidente, ministra Calderone, la sicurezza sul lavoro è un tema importante e di attualità perché purtroppo ogni giorno si perdono tre vite. Anche la scuola è un luogo di lavoro, non solo di apprendimento, dove il personale scolastico deve essere tutelato, ma anche gli stessi allievi nella loro salute e sicurezza, nelle attività extra scolastiche, nei tirocini e nelle attività di apprendistato. Storicamente la tutela assicurativa in ambito scolastico era limitata allo svolgimento di esperienze esperienze tecnico scientifiche ed esercitazioni nonché all'uso non occasionale di alcune tipologie di macchinari. L'articolo 18 del decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48, voluto prontamente da questo Governo, ha stabilito l'estensione per l'anno scolastico 2023-2024 dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro ai settori dell'istruzione, della formazione e anche alla formazione aziendale. Chiedo quindi al signor Ministro, tramite lei, Presidente, quali siano stati gli effetti ottenuti a seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL al comparto scuola e come

sociali*. Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti per aver voluto affrontare un tema estremamente importante. Il Governo considera la protezione dei nostri studenti una priorità assoluta, consapevole che la scuola rappresenta un luogo centrale per la crescita e la formazione delle nuove generazioni. Garantire un ambiente sicuro e protetto è essenziale non solo per l'apprendimento, ma anche per il benessere complessivo degli studenti e di tutto il personale scolastico. n. 48, ha segnato una svolta importante, estendendo per l'anno scolastico e accademico 2023-2024 l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL al mondo della scuola. Non è un intervento soltanto tecnico, ma rappresenta un impegno concreto del Governo per tutelare tutti coloro che partecipano alle attività didattiche, dai docenti agli studenti, garantendo loro copertura assicurativa anche in contesti educativi prima non contemplati. I primi risultati di questa estensione sono estremamente incoraggianti. Il numero di soggetti assicurati è cresciuto in modo significativo, permettendo di coprire incidenti e infortuni in settori che prima non godevano di queste protezioni. Significa che sempre più studenti e lavoratori del settore scolastico possono contare su un sistema di sicurezza più ampio e inclusivo. Gli ultimi dati INAIL sull'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali risentono degli effetti dell'estensione assicurativa operata con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, la cui efficacia è raccontata dai dati relativi agli ultimi tre anni scolastici, dunque rilevati tra il 1° settembre e il 30 giugno. In particolare, si osserva come le denunce di infortuni degli studenti siano passate dalle 60.244 dell'anno scolastico 2021-2022 alle 75.290 dell'anno scolastico 2023-2024, facendo registrare un incremento cento (uguale per studenti e studentesse), il che testimonia l'efficacia della copertura. Contestualmente all'incremento delle denunce di infortunio degli studenti c'è stato anche un significativo incremento delle definizioni positive, passate da 28.888 dell'anno scolastico 2021-2022 alle 48.902 dell'anno scolastico 2023-2024. Questi dati hanno sostenuto il nostro impegno a rinnovare la copertura assicurativa anche per l'anno scolastico da poco cominciato. Vogliamo dare continuità a questa misura, individuando al contempo percorsi e risorse per attivare ulteriori interventi a tutela della sicurezza in ambito scolastico. I giovani sono il nostro futuro e il futuro dell'Italia ed è nostro dovere proteggere la loro salute e rendere sicuri i luoghi in cui si formano. In questi due anni abbiamo realizzato numerose attività con le scuole per coinvolgere attivamente gli studenti sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e abbiamo riscontrato una sensibilità un'attenzione sorprendenti. Sono certa che, con l'impegno di tutti, riusciremo a diffondere la cultura del lavoro sicuro e garantisco al Senato che il Governo proseguirà sul percorso sino ad oggi tracciato.

di vita per gli alunni e ambiente di lavoro per gli insegnanti; è il luogo primario della prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell'individuo e del gruppo fin dai primi momenti della socializzazione. L'educazione scolastica è infatti determinante nell'impostare negli individui comportamenti adeguati agli stili di vita sani, oltre che nel favorire l'interlocuzione delle regole e dei valori fondamentali di responsabilità sociale e civile. Di fronte all'incremento del tasso di mortalità e malattia dovuto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, è fondamentale rivalutare rivalutare il ruolo educativo e formativo della scuola nel fornire gli strumenti culturali e le competenze relazionali utili all'inserimento in una futura realtà lavorativa. È quindi importante quello che sta facendo questo Governo per inserire nei percorsi formativi la sicurezza sul lavoro e per investire - come lei ha confermato

come lei sa da tempo si discute del fatto che abbiamo, dentro il mondo del lavoro, una crescita del lavoro povero, che è in difficoltà a mantenere la propria condizione di autosufficienza, che dovrebbe essere la prima condizione e il primo esito del lavoro. Eppure, come sappiamo, rispetto a questo è stata spesso usata la categoria degli occupabili, che avete ampiamente utilizzato nella cosiddetta

effetti di quella che è stata poi definita SFL, cioè l'attivazione dei percorsi di formazione e lavoro, affinché quegli occupabili diventassero effettivamente componenti del mondo del lavoro. Gli ultimi dati noti provengono da un report dell'INPS, i cui numeri tutto sommato non tornano, perché parrebbe che dell'SFL hanno beneficiato solo 140.000 lavoratori. che vi era una platea potenziale prevista di 436.000 lavoratori. La prima domanda che ci viene in mente è cosa sia successo di tutti questi. questi. Ci risultainoltre che siano circa 30.000 le persone che hanno trovato un lavoro attraverso il sistema informativo che è stato attivato e che, peraltro, è stato ulteriormente implementato dal fatto che su quella piattaforma vi sono anche i lavoratori in disoccupazione, in cassa Le domande che vorrei porle dipendono da un tema che credo dovrebbe vedere tutto il sistema lavorare congiuntamente. La formazione è uno degli elementi fondamentali per il mercato del lavoro. cosa vorrei sapere: quali sono davvero le persone cosiddette occupabili, ex percettori di reddito, che hanno effettivamente trovato lavoro. Inoltre, quanti sono i progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale che derivano dal decreto-legge n. 48 del 2023 che siano stati effettivamente attivati; infine, cosa si intende fare per migliorare e rendere efficiente il sistema delle politiche attive e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Perché se dobbiamo basarci sui numeri a cui facevo 30.000 persone a fronte di 300.000 potenziali posti di lavoro, evidentemente il sistema non dà le risposte che sono necessarie. PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, dottoressa Calderone, ha Signor Presidente, ci vorrebbe molto tempo per poter dare una risposta esaustiva con tutti i dati che sono stati richiesti, ma cercherò di essere breve. Con riferimento all'interrogazione illustrata, segnalo che i dati richiesti sono rinvenibili consultando l'osservatorio INPS sulle misure dell'assegno di inclusione e del supporto per formazione e lavoro. Sul punto sono state accolte quasi 700.000 domande relative all'assegno di inclusione che fanno riferimento ad altrettanti nuclei familiari e che coinvolgono circa 1,7 milioni di cittadini: il *target* della platea che era stata ipotizzata in legge di bilancio. Per quanto riguarda il supporto per la formazione e il lavoro, sono state 96.000 le persone a cui è stata accolta la domanda ed erogata la prestazione. Il periodo di riferimento va dal primo mese di operatività della misura (settembre 2024 per l'assegno di inclusione) e, per i pagamenti, fino a maggio 2024 (ultimo mese in cui i dati possono ritenersi statisticamente consolidati). In particolare a maggio 2024 il numero di nuclei beneficiari dell'assegno di inclusione è stato pari a 625.000, mentre l'importo medio erogato mensilmente è pari a 617 euro. Per quanto riguarda il supporto per la formazione e il lavoro, i beneficiari tra settembre e dicembre 2023 erano 33.000, aumentando a 93.000 tra gennaio e maggio 2024. Complessivamente, le domande accolte fino a giugno 2024 sono state 96.000. Con riferimento alla platea degli ex percettori di reddito di cittadinanza, a partire dal 1° gennaio 2023 a tutt'oggi hanno avuto almeno un rapporto di lavoro nel periodo circa 500.000 soggetti. Ovviamente la lettura di questo dato può innescare una serie di riflessioni: una fra tutte è la valutazione degli impatti sul supporto per formazione e lavoro (SFL). Se consideriamo che molti dei fruitori hanno comunque dei rapporti di lavoro sia pur temporanei con bassa retribuzione, è anche ragionevole che la platea già impiegata a vario titolo non abbia fatto domanda per per SFL. I soggetti che invece hanno trovato lavoro dopo la sottoscrizione del piano di attivazione digitale (PAD) sono 26.845. È utile segnalare che sul sistema di inclusione sociale e lavorativa sono presenti 27.303 corsi di formazione, pari a 419.727 posti, mentre sono attivi ad oggi 5.957 progetti utili collettività, per complessivi 75.569 posti. Ricordo che il supporto per la formazione e il lavoro nasce per ripristinare il criterio di attivazione e e condizionalità nelle politiche attive. Il *target* di riferimento era un *target* potenziale che si è notevolmente ridotto a causa dell'andamento dell'occupazione che, come è noto, ha raggiunto il *record* più alto degli ultimi vent'anni. In questo contesto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a creare il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, che consente l'attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa. Nel suo sviluppo, la piattaforma ha già l'obiettivo di favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro, peraltro erogando numerosi servizi a livello Da ultimo, rappresento che, già dal mese di novembre, come previsto dal decreto legge coesione, verranno utilizzati tutti i dati dei beneficiari di Naspi e Dis-Coll in collaborazione con tutti i Centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro presenti in piattaforma, fornendo un nuovo e importante servizio al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in maniera efficiente e sistematica. Voglio ribadire, in ultimo, che la piattaforma che è stata creata non è solo ed esclusivamente rivolta a a fornire servizi e a erogare prestazioni agli ex percettori di reddito di cittadinanza, oggi titolari di assegno di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. È rivolta a questi soggetti, ma è ancor più rivolta a tutti coloro i quali, in Italia, cercano lavoro e vogliono cambiare lavoro.

pur avendo fornito molti numeri rispetto alle azioni che avete deciso di intraprendere, che sono tutte però azioni che spezzettano le platee di riferimento e quindi non danno risposte universali alle persone, il punto fondamentale continua ad essere quello di quali politiche facciamo per l'occupabilità non di chi è già nel mercato del lavoro ed è in grado di agire concretamente, ma di quelle persone che ne sono in qualche modo estranee. La preoccupazione è sui numeri che non tornano mai, perché si perdono nel nulla, ma evidentemente sono persone che stanno nel nostro Paese, che esistono e che avrebbero bisogno delle risposte. In realtà, continuare a disgregare e a perdere di vista gli strumenti permette la crescita di un lavoro sommerso e irregolare, la scomparsa delle persone e quindi una condizione negativa. Credo che non si possa cancellare questo dato dicendo che l'occupazione intanto è aumentata, perché vorrei ricordarle, Ministro - lei lo sa benissimo - che giusto nel rapporto INPS di qualche giorno fa un milione di persone risulta avere una settimana contributiva nell'anno. Allora, capisco che sono sicuramente state occupate, ma non sono certamente persone in condizioni di gestire autonomamente la loro vita e che si possono considerare

la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce un'assoluta priorità di cui le istituzioni sono chiamate a farsi carico, in quanto ogni infortunio mortale sul lavoro rappresenta una profonda ferita per l'intera società; i dati pubblicati da INAIL il 3 settembre 2024 rilevano come, rapportando il numero dei casi di infortuni mortali agli occupati ISTAT, nel confronto tra i primi sette mesi del 2019 (ultimo anno pre pandemia) e lo stesso periodo del 2024, l'incidenza scenda da 2,59 decessi denunciati

tramite interventi legislativi mirati ed efficaci. In tale scenario, il decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2024 ha previsto, all'articolo 29, l'introduzione l'introduzione dal 1° ottobre nel 2024 della patente a crediti per l'edilizia, dando finalmente attuazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2009, che prevedeva un sistema di qualificazione delle imprese. In attuazione alla suddetta disposizione, il 20 settembre 2024 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, che va proprio a regolare le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei temporanei o mobili. Si chiede quindi di sapere quali siano i punti di forza del nuovo sistema di qualificazione delle imprese e come si ritenga che la patente a crediti possa incidere sulla prevenzione e il contrasto degli infortuni sul lavoro.

come si diceva, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese: la cosiddetta patente a crediti: una misura senza precedenti che risponde, allo stesso tempo, una richiesta storica che veniva dalle parti sociali di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008. La tutela della sicurezza sui luoghi del lavoro e la promozione della cultura della prevenzione sono al centro del programma di Governo e ne hanno caratterizzato l'azione sin dall'insediamento. D'altronde, proprio come indicato da quest'Assemblea con una mozione unitaria, è nostra responsabilità garantire che ogni lavoratore operi in condizioni di sicurezza adeguate, in particolare nei settori più a rischio. In questo senso, il sistema di qualificazione delle imprese basato su crediti sarà operativo a partire dal 1° ottobre 2024, con possibilità di presentare la relativa domanda sull'apposito applicativo reso disponibile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente a crediti offrirà una dotazione iniziale di 30 crediti alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri, con la possibilità di ottenere ulteriori crediti sulla base di altri criteri, come lo storico aziendale e l'assenza di provvedimenti di decurtazione, la partecipazione a percorsi formativi specifici, l'avvio di di investimenti mirati. Il meccanismo di assegnazione e di eventuale penalizzazione è regolato, come si ricordava, dal decreto ministeriale 18 settembre 2024, Inoltre, per dare alle imprese modo di operare immediatamente, già dal 1° ottobre è possibile presentare via PEC una dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. Quella della patente a crediti una misura ambiziosa, le cui prospettive sono di grande impatto. Implementiamo il sistema di sicurezza nei cantieri, incentivando le imprese a mettere in atto le migliori pratiche in materia di sicurezza che garantiscono una graduale riduzione degli incidenti sul lavoro, e valorizziamo chi adotta pratiche virtuose secondo un principio di responsabilità progressiva dato dal riconoscimento dei crediti, favorendo lo sviluppo di azioni concrete sul piano della prevenzione della formazione e degli investimenti. È la cifra del nostro agire da quando ci siamo insediati come Governo: promuovere a tutti i livelli la cultura della prevenzione. Oltretutto, la patente ci consentirà di creare un sistema di maggiore trasparenza che permetterà di identificare più chiaramente le imprese che operano in conformità con gli *standard* di sicurezza, aumentando così la fiducia nei confronti degli operatori del settore. È proprio per questo che ritengo sia essenziale, a questo fine, un'azione concertata con il coinvolgimento di imprese e lavoratori. Per questo, abbiamo attivato una campagna informativa capillare per chiarire i dettagli applicativi della misura, promuovendo *webinar*, incontri e tavoli di confronto con le principali associazioni di categoria e i sindacati. In conclusione, la patente a crediti rappresenta una misura innovativa oggi rivolta al mondo dell'edilizia, ma estendibile in futuro ad altri settori, che potrà portare benefici tangibili in termini di sicurezza sul lavoro e competitività delle imprese. In questo senso sarà determinante la collaborazione delle parti sociali, cui rivolgo il mio invito affinché, come avvenuto in tutta la fase di elaborazione della misura, si riesca a giungere uniti all'obiettivo comune di assicurare ai lavoratori contesti del lavoro sempre più sicuri e tutelati.

Presidente, voglio ricordare in quest'Aula Massimo Canalini, un nome oggi forse sconosciuto ai più, ma che ha lasciato un segno importante. Dalla sua città, Ancona, nel decennio tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, Canalini ha sperimentato il crocevia di una nuova scena letteraria. Massimo Canalini ha rivoluzionato

Pier Vittorio Tondelli fu bruciante e stellare e diede vita ad una delle esperienze più dirompenti per la nostra cultura, cambiando nel profondo non solo la narrativa, ma l'intero immaginario collettivo di un Paese, il nostro, in profondissima trasformazione. Irruppero voci nuove e urgenti, bisogni esistenziali, periferie e linguaggi che reclamavano spazio. In Ancona, Canalini aveva fondato con Giorgio Mangani «Il lavoro editoriale» e poi diede vita alla leggendaria "Transeuropa", molto più di una casa editrice, un laboratorio che ruppe canoni e convenzioni, chiamando a raccolta una nuova generazione: Enrico Brizzi, Silvia Ballestra, Angelo Ferracuti, solo per fare qualche nome. Egli convinse Joyce Lussu a pubblicare con "Transeuropa" uno dei suoi libri più belli - «Portrait» -, il romanzo di una vita per immagini. Signora Presidente, ho di Massimo Canalini dei ricordi personali che dicono molto di lui e ai quali tengo molto. All'inizio di settembre del 1999, durante il secondo dei nostri anni anconetani, con mia moglie Cristina prendemmo una casa in affitto in via Goito, la strada che da piazza Roma si arrampica come una vertigine verso il faro; era all'ultimo piano, poco più di un monolocale, freddo e umido, ma con intorno una terrazza bellissima, da cui si vedeva tutta Ancona fino al porto e al mare. Al piano terra di quella palazzina di inizio Novecento abitava Canalini con la sua giovane compagna, Alessia. Un giorno lo vidi che, sporgendosi da una finestra che quasi toccava terra, simulava un gesto teatrale, di eroismo o di protesta o non so. Ci conoscemmo in quella comune militanza di affittuari. Mia moglie e la sua compagna divennero molto amiche, anche perché entrambe incinte. Il nostro primo figlio, Federico, e il loro figlio, Pier Vittorio, nacquero negli stessi giorni. Una volta, a casa sua in quel pianterreno, mentre discutevamo animatamente, Massimo troncò tutto e disse che comunque la cosa più importante era il rock. E lì, seduta stante, mi regalò il suo disco preferito dei Led Zeppelin, quello con all'interno la canzone «Stairway to heaven». E allora ci abbracciammo, sotto gli sguardi attoniti e un po' straniti di Alessia, di Cristina, dei piccoli Pier Vittorio e Federico. Furono anni belli e romantici. E questo fu anche Massimo Canalini. *(Applausi)*.

trovo del tutto fuori luogo le risate con cui il ministro Calderoli, ieri, in occasione di un'audizione tenutasi presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha accolto alcune domande da me poste.

criteri determinati sulla base delle caratteristiche dei territori, del clima, del costo della vita e della demografia. Analizzando questi parametri, onorevoli colleghi, riflettiamo tutti su cosa significano: da un punto di vista razionale, equivalgono a legittimare una differenziazione dei diritti sulla base del criterio di nascita,

Siamo intellettualmente onesti, però: questo evidenzia la logica secessionista secondo cui, laddove c'è maggiore ricchezza, ci devono essere anche migliori servizi e ulteriori diritti. L'aspetto più grave è che noi parlamentari non possiamo mettere bocca su queste metodologie elaborate dai tecnici del CLEP, presieduto dal noto giurista Sabino Cassese. Chi sono questi tecnici? Ne cito alcuni: l'onorevole Marco Stradiotto, che lavora da tempo al federalismo fiscale; la presidente Elena D'Orlando, storica consulente del leghista Zaia; il professor Andrea Giovanardi, già consulente della Regione Veneto; il professor Giovanni Guzzetta, consulente della Regione Lombardia. Ho fatto richiesta al Ministro - richiesta sacrosanta - che il lavoro effettuato dagli esperti venga sottoposto al voto parlamentare e inoltre ho esortato a rendere pubblici i verbali delle riunioni del CLEP e gli ho chiesto dove fossero le risorse per finanziare i LEP, che, secondo molti giuristi, ammontano ad oltre 100 miliardi. Purtroppo, reputo a dir poco imbarazzante l'atteggiamento del ministro Calderoli, anzi tengo a precisare che si è limitato a leggere una relazione sicuramente prodotta dalla Commissione tecnica

Onorevoli colleghi, questo atteggiamento non ha mortificato tanto la mia figura e quella di tutti gli altri parlamentari, quanto tutte le istituzioni e, soprattutto, milioni di italiani.